Presidente, la vicenda collegata alla morte di Giuseppe Uva è da molto tempo all'attenzione degli uffici del mio Ministero. Si tratta di una vicenda particolarmente dolorosa, tutt'ora con dei punti oscuri che devono essere chiariti e rispetto ai quali non si è ancora pervenuti a una risposta giudiziaria convincente. Come sapete, proprio per questa ragione, di recente ho ritenuto di ricevere personalmente i familiari del signor Uva per ribadire loro la mia personale vicinanza e il mio impegno nella ricerca della verità. Sul piano istituzionale, vi informo che, sin dalle prime segnalazioni ricevute dagli uffici ministeriali, sono state tempestivamente intraprese tutte le iniziative conoscitive e ispettive volte ad accertare la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare in capo ai magistrati che, a diverso titolo, si sono occupati della vicenda. I risultati sono stati negativi, e anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione, titolare anche egli dell'azione disciplinare, ha escluso la sussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, con ciò procedendo all'archiviazione degli atti in data 9 maggio 2011 e 13 dicembre 2012. Devo però subito aggiungere che successivamente, nell'ambito del procedimento penale della procura di Varese conseguente alla trasmissione degli atti al pubblico Ministero, disposta dal tribunale di Varese con sentenza del 23 aprile 2012, con la quale si indicava la necessità di approfondimenti investigativi su quanto era accaduto prima del ricovero in ospedale dell'Uva, il giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza in camera di consiglio, a seguito dell'opposizione delle parti offese alla richiesta di archiviazione formalizzata dal pubblico ministero con riguardo alla posizione processuale di coloro che si trovavano nella caserma dei Carabinieri di Varese, ove il predetto Uva era stato condotto subito dopo il fermo di identificazione della polizia giudiziaria. Il tema di indagine da approfondire (l'udienza sarà tenuta dal giudice il prossimo 8 ottobre) è quello dell'accertamento dei fatti accaduti prima dell'ingresso dell'Uva in ospedale, nonché della provenienza e della valenza causale dei traumi rilevati sul corpo del predetto che, secondo il giudice, avrebbero rappresentato una possibile concausa del decesso. Si tratta di un fatto processuale di grande rilevanza - in particolare per le censure di merito che il giudice ha rassegnato in ordine all'attività investigativa - che richiede un esame approfondito da parte degli uffici competenti perché potenzialmente idoneo a far luce sulle effettive responsabilità

confermo di aver dato incarico alle competenti articolazioni ministeriali, ed in particolare all'ispettorato generale, affinché acquisiscano tutti gli elementi conoscitivi necessari a far luce sull'intera vicenda. A questo posso solo aggiungere, data la delicatezza degli accertamenti, che il procuratore generale presso la corte di appello di Milano e il presidente del tribunale di Varese hanno già trasmesso all'ispettorato generale informazioni ed atti che saranno utili per lo svolgimento delle verifiche delegate. Altri atti dovranno ancora essere trasmessi dalla procura della Repubblica di Varese. In ogni caso, occorrerà naturalmente attendere l'esito dell'udienza camerale sopra indicata, anche al fine di verificarne l'incidenza su fatti e circostanze di possibile rilievo disciplinare. Concludo, infine, rassicurando gli interroganti che gli accertamenti e gli esami si stanno svolgendo con il massimo impegno e con la dovuta celerità, in modo da consentirmi di assumere, nel più breve tempo possibile - compatibilmente con la loro complessità - le mie eventuali determinazioni sul piano disciplinare.

mi dichiaro parzialmente soddisfatto e spiego immediatamente il senso di questa mia affermazione. Io la ringrazio molto e sentitamente per la rapidità,

e sullo sfondo c'è la questione di ciò che costituisce fondamento stesso dello Stato di diritto, ovvero il suo dovere di tutelare l'integrità e l'incolumità di quanti sono affidati alla sua custodia. Ciò non è avvenuto nel caso di Giuseppe Uva.

si possa avviare un'indagine che porti ad accertare quanto avvenne in quel tempo e in quello spazio (le quasi tre ore trascorse da Giuseppe Uva nella caserma dei carabinieri di Varese),

di Varese. Noi tutti ci auguriamo che, con l'udienza dell'8 ottobre, prima che la prescrizione giunga a cancellare questa atroce vicenda, la ricerca della verità e della giustizia possa essere avviata, ricordando che se questo percorso inizia solo ora e con tanto ritardo lo si deve - e questa responsabilità non può essere ignorata e va tutta accertata - anche alla ostinata, pervicace negligenza di un pubblico ministero che per cinque anni non ha fatto ciò che poteva e doveva.

Grazie, signor Presidente. e di fornire la conseguente quantificazione del fabbisogno economico necessario a garantire totale copertura alla salvaguardia di tali lavoratori. In via preliminare, si ritiene opportuno precisare la distinzione, già in più occasioni esposta dal ministro Giovannini, tra i lavoratori cosiddetti esodati e quelli cosiddetti bloccati. I primi sono coloro che risultano espulsi dal sistema produttivo e sono bisognosi di misure di salvaguardia in termini di requisiti pensionistici e di accompagnamento alla pensione, qualora gli strumenti di sostegno al reddito non consentano di garantire loro una tutela anche minima, fino al raggiungimento del diritto a pensione entro un termine ragionevole (generalmente 24-48 mesi). I secondi sono quei lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione ma non ancora espulsi dal mercato del lavoro. I cosiddetti esodati, quindi, sono soggetti già espulsi dal mercato del lavoro prima della riforma pensionistica del 2011, i quali, per effetto dell'innalzamento dei requisiti per il conseguimento a pensione (anzianità o vecchiaia), non raggiungono entro un limite ragionevole tale diritto. Peraltro, cosa di non poco conto, questi lavoratori appartengono a categorie piuttosto circoscritte, censite ed identificate dall'INPS (disoccupati, cassaintegrati, lavoratori in mobilità o cessati a pochi mesi dall'età di pensionamento), la stima dei relativi contingenti numerici non pone eccessive difficoltà pratiche. Al riguardo, occorre precisare che il ministro Giovannini, quando il 16 maggio 2013 intervenne in quest'Aula sul problema che oggi torna all'attenzione dell'Assemblea, aveva già chiesto ed ottenuto da alcuni giorni (l'8 maggio) che l'INPS fornisse una fotografia esatta dello stato dell'arte, corredata da precisi dati numerici relativi allo stato delle lavorazioni riferite a ciascuna delle platee delle tre tornate di salvaguardia varate fino a quel momento. Ciò rappresenta una conferma dell'atteggiamento di trasparenza e di piena collaborazione con il Parlamento che ha caratterizzato fin dall'inizio l'operato del Governo in carica su questo delicato tema. Diverso è il caso dei cosiddetti lavoratori bloccati. Il problema di tali lavoratori, infatti, rappresenta più in generale un problema del sistema produttivo e delle sue prospettive occupazionali, nel senso che l'innalzamento repentino dei requisiti pensionistici, in particolare quelli di anzianità, ha limitato o eliminato lo strumento principale finora utilizzato per le ristrutturazioni aziendali,

i programmi di ristrutturazione aziendale abbiano durata pluriennale (è il caso degli accordi per la mobilità che prevedono cessazioni dal lavoro negli anni futuri, Pertanto, in merito all'individuazione e alla quantificazione dei soggetti, non può che farsi riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme. È però importante sottolineare che la difficoltà di quantificare il numero dei lavoratori cosiddetti bloccati non deriva da un atteggiamento inerte o negligente da parte del Governo, ma costituisce una conseguenza diretta del fatto che il fenomeno in questione rappresenta una variabile dipendente da fattori economici e produttivi e da scelte individuali di lavoratori ancora attivi in continuo divenire, che non sempre si riesce ad individuare con precisione mancando le informazioni necessarie. Passo ora a fornire alcuni dati numerici relativi allo stato di attuazione delle tre tornate di salvaguardia

la platea dei salvaguardati è stata inizialmente stimata in 65.000 soggetti in possesso dei requisiti indicati nel decreto interministeriale in data 1° giugno 2012

Con il decreto-legge n. 95 del 2012, denominato *spending review*, si è poi aumentato di ulteriori 55.000 unità il numero dei salvaguardati

secondo una progressione di spesa che prevede stanziamenti di risorse fino al 2020 (tutto il periodo che intercorrerà fino a che questi lavoratori matureranno il diritto alla pensione). Il decreto ministeriale 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013,

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le cui modalità di utilizzo saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. la cui dotazione per l'anno 2013 ammonta a 36 milioni di euro - confluiranno anche le eventuali economie accertate a consuntivo ed aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei decreti interministeriali del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013: in altre parole, tutti i decreti che hanno previsto la salvaguardia delle varie tornate potranno produrre delle economie, che andranno a confluire nel fondo. In tal modo verrà assicurata una ridestinazione stabile nel tempo delle risorse finanziarie appostate ai fini della risoluzione del problema dei salvaguardati, con integrale riutilizzo degli eventuali risparmi per le medesime finalità. Nel contempo, si precisa che sono state avviate le attività di liquidazione delle prime pensioni ma l'impegno del Governo a fornire una risposta credibile e strutturale al problema richiamato dalla senatrice interrogante non può certo dirsi esaurito e, anzi, proprio in questi giorni si è concretato in un ulteriore risultato tangibile: la quarta salvaguardia. Infatti, il decreto-legge n. 102 del 2013, adottato lo scorso 31 agosto (il cosiddetto decreto IMU-CIG in deroga), interviene a sostegno dei lavoratori cosiddetti licenziati individuali (un'ulteriore categoria che si aggiunge alle precedenti), Gli esodati si allargano, infatti, come numero sulla base dell'individuazione di categorie alle quali viene riconosciuto il diritto di andare in pensione con le precedenti regole

alle precedenti), i quali hanno interrotto il proprio rapporto prima dell'applicazione della riforma sulle pensioni e che, per effetto di essa, si sono trovati al contempo privi di stipendio e di pensione. quarta salvaguardia - dall'applicazione della riforma del 2011 viene così ulteriormente incrementata di 6.500 unità. In definitiva, si conferma che la questione segnalata interrogante riveste assoluta centralità per l'Esecutivo e per il Ministero del lavoro in quanto coinvolge interessi e valori vitali per l'individuo ed evidenzia una situazione di forte disagio, tuttora presente, e di allarme sociale,

Come dico sempre, avere i soldi per poter andare avanti serve a dare speranza e a crearsi una prospettiva,

lei, Sottosegretario, crede di vedere solo me e la collega Moronese qui davanti a lei, ma c'è tutta una Regione, e le voglio dire che è la forza di tutta questa gente, anche di quella che non ci ha votato, che ci ha spinto fin qui di fronte a lei. Non ricordiamo un'altra ragione Quindi la preghiamo di ascoltarci con molta attenzione perché è la Campania che le parla. Da oltre vent'anni nella nostra area, compresa tra il litorale domizio-flegreo, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano-vesuviano e la città di Napoli, si consuma un delitto. Ma «delitto» è una parola insufficiente: bisognerebbe parlare di strage ambientale, perché lo sversamento continuo di rifiuti speciali e tossici, dati alle fiamme ogni giorno, più volte al giorno, colpisce le persone, ma colpisce tutto un ecosistema, l'aria, la terra e l'acqua; compromette irrimediabilmente un intero territorio e la sua stessa speranza di vita; colpisce al cuore la sua economia condannandola al disastro ambientale e sociale. Basterebbero le troppo numerose foto che ogni giorno vengono diffuse in rete dalle centinaia di cittadini che abitano questa vasta area delle province di Napoli e Caserta, nota come la «terra dei fuochi», per avere un'idea chiara del dramma ambientale che affligge questo territorio. Vorrei poterle mostrare quelle foto e farle vedere i video, farle leggere le innumerevoli denunce inascoltate, lettera morta da decenni. farle sentire le registrazioni delle telefonate di denuncia alle forze dell'ordine, che declinano l'invito ad intervenire adducendo giustificazioni come la mancanza di personale e mezzi (auto e benzina). L'appuntato Giovanni Parascandola, come emerso dal processo «Rompiballe», metteva la benzina di tasca propria per fare le indagini e smuovere chi di dovere. Le forze dell'ordine forniscono altri numeri di telefono perché la cosa non è di loro competenza o attaccano senza più rispondere, perché indifferenti o forse inermi e sconfitti. vorrei poterla accompagnare su quei territori, come abbiamo fatto due mesi fa con i nostri colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma so che lei è al corrente di questi fatti, così come è al corrente e al lavoro il suo Ministero. Quello che vogliamo però qui sottolineare è l'imponenza dell'impianto economico-industriale che sta all'origine di questo fenomeno. È quantomeno insufficiente indagare solo nella bassa delinquenza locale e nella rete di attività commerciali in nero che producono principalmente borse e scarpe, come sta facendo il commissario ai roghi tossici Cafagna. Non basta. Bisogna capire che siamo di fronte alla più grande organizzazione industriale ed economica di questo Paese, ad uno scellerato progetto di dimensioni colossali, che muove miliardi di euro ed interessi da oltre vent'anni: ce lo ha ricordato Schiavone in questi giorni. Il vero colosso industriale italiano è questo, con un fatturato molto maggiore di quello del traffico di droga: lo smaltimento a basso costo di enormi quantità di rifiuti industriali e tossico-nocivi provenienti da tutte le Regioni d'Italia, e forse anche dall'Europa. Questo fenomeno è stato indagato più volte dalla magistratura in innumerevoli processi, come il processo «Cassiopea», finito in prescrizione appena due anni fa. Eppure il meccanismo è semplice, è registrato dalle telecamere ed è evidente: una montagna più alta del Gran Sasso che manca all'appello dei rifiuti industriali. Siamo disponibili ad affrontare questo colosso industriale e a sconfiggerlo? Agli atti leggiamo: «Partivano da Milano, Vicenza, Padova, Treviso, Verona, Venezia, Bergamo e Brescia, con una regolarità di circa cento viaggi a settimana, per essere sversati nelle campagne campane. I camion trasportavano fusti che contenevano polvere residuata dall'abbattimento dei fumi delle industrie siderurgiche e metallurgiche, oli minerali, lubrificanti delle macchine, scarti delle vernici, ceneri residue da combustione, solventi, acque provenienti da stabilimenti di industrie chimiche e acidi. Appena arrivavano in Campania venivano sepolti nelle campagne coltivate, lungo le strade sterrate, in terreni comprati da contadini indebitati o spesso nemmeno comprati, semplicemente si pagava una tangente che lasciava sversare nella propria terra, stipati in discariche legali dove finivano i rifiuti cittadini, in quelle abusive, nelle cave». Forse la crisi economica e i riflettori hanno smorzato un poco il traffico, ma questo continua. O si mette al centro questo e si risolve o non si è risolve niente. O si capisce che non è un problema locale, regionale, ma un problema nazionale (invece di sottrarre i territori ai SIN) o non si è capito niente. Sconcertano le affermazioni di Cafagna in prefettura la primavera scorsa che alla presenza del ministro Orlando, nel fare la sua relazione di aggiornamento, si sofferma sul «lancio del sacchetto tanto in voga da queste parti, a cura di gente che preferisce darsi a questo *sport* piuttosto che affidarsi al servizio di raccolta differenziata offerto offerto dalle amministrazioni locali». Nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta del 5 febbraio 2013 - ossia ieri - si legge: «Deve osservarsi come nessuna attività efficace sia stata messa in atto. È possibile tamponare i singoli episodi, ma non il fenomeno, che continua a persistere». Ecco, ci sembra che finora con le azioni messe in atto con il commissariamento dal novembre scorso si sia continuato a fare solo questo: tamponare singoli episodi, ma non il fenomeno, che continua a persistere. Apprezziamo però molto l'interessamento del ministro Orlando alla questione e gli riconosciamo un approccio diverso, una volontà di rendere più strutturale l'azione,il fatto stesso che sia intervenuto sulla *gaffe* della ministra Lorenzin e ne abbia corretto il tiro. il tiro. Tanti operatori mi sollecitano a chiedere che siano messi a sistema e resi fruibili e noti i risultati delle schede di dismissione ospedaliera (SDO), al fine di venire a conoscenza per semplice interpolazione della situazione di salute di ogni territorio, e invece si continua da decenni a parlare del registro tumori registro tumori mentre i dati già li abbiamo. Lo studio ARPAC-AMRA 2010 ha evidenziato: inquinamento diffuso delle falde indagate; contaminazione dei suoli, per cui è necessario procedere all'analisi del rischio; presenza di superamenti *hot spot* di diossine e furani alla presenza di rifiuti combusti. Studi ed analisi dei dati sanitari relativi alle percentuali di malattie tumorali riscontrate nei territori coinvolti, condotti dall'Istituto superiore di sanità, dalla fondazione Pascale, dall'università Federico II e dalla stessa procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno evidenziato un aumento indiscusso di patologie tumorali. In soli dieci anni, i decessi per tumore sono incrementati del 47 per cento. I dati raccolti dall'istituto Pascale di Napoli hanno evidenziato che il tasso di mortalità femminile per tumore al polmone è il più alto in Italia, con un aumento del 100 per cento

Dal documento di sintesi della ricerca epidemiologica condotta in Campania dall'ISS è emerso che per quanto riguarda i tumori maligni nel loro complesso, la mortalità in Campania è superiore ai valori dell'intera Italia per il contributo delle province di Caserta e di Napoli. Condividiamo - come abbiamo detto - la volontà del ministro Orlando di procedere diversamente, ad esempio di coinvolgere il Ministro dell'agricoltura in tale questione al fine di creare una mappatura dei territorio che sia nota e certa, con certificazioni di qualità per le aree sane che producono una sana economia agroalimentare, che va salvaguardata anche dalla cattiva notorietà dei luoghi, fermando al contempo ogni attività di coltivazione e pascolo laddove sia accertato lo stato di compromissione ambientale: ma quando? Ci troviamo ancora concordi con il Ministro nella volontà di inasprire i reati ambientali superando il salvacondotto della prescrizione e di voler procedere con il sequestro dei beni per risanare e non per risarcire il danno. La nostra volontà è ben espressa nella proposta di legge Micillo presentata Ci piace, ancora, l'azione concreta di chiudere al traffico di rifiuti in entrata in Campania, ma ci chiediamo a cosa servirà se questo è previsto per soli due anni. Siamo ancora compiaciuti nell'apprendere che il SISTRI, dopo aver depotenziato il sistema MUD, creato difficoltà, vuoti, incertezze

Internet «Prometeo», che si poneva l'obiettivo di raggiungere la popolazione in un rapporto diretto, trasparente e continuo, non racconta niente, si raggiunge solo dal sito della prefettura di Caserta, non è un sito facilmente fruibile (invito i più a dirmi se lo conoscono), mentre tutti conoscono, ahimè, il sito la «Terra dei Fuochi» che, al contrario di «Prometeo», non è costato niente alla collettività. Sul sito leggiamo che i roghi sono dimezzati nel semestre 2013 rispetto al semestre 2012, ma come e dove purtroppo alla gente non risulta, le denunce continuano e la situazione sembra assolutamente invariata. Se sono dimezzati i fuochi, a fronte di quanti arresti effettuati e quante attività illecite fermate? Leggiamo sul sito che è stato compiuto un arresto, un'attività è stata fermata. Noi stessi stiamo lavorando a un disegno di legge che istituisca un organismo nazionale che coordini le indagini relative alla criminalità organizzata in ambito ambientale, sul modello dell'organigramma

Anche il patto per la «terra dei fuochi», concluso con i vari Comuni, ci sembra un ottimo documento, un bel pezzo di carta, un buon progetto di riorganizzazione territoriale, ma dove sono gli adeguati fondi, gli uomini, i mezzi e le forze? Come avverrà tutto questo e, soprattutto, quando? Ecco perché, Sottosegretario, le poniamo le domande di questa interpellanza, che sono Grazie,

Con riferimento alle problematiche ambientali segnalate dagli interroganti con l'interpellanza n. 42, è utile premettere che l'illegale smaltimento di rifiuti e l'accensione di roghi di materiale spesso tossico nei territori delle province di Napoli e Caserta

Il fenomeno cosiddetto terra dei fuochi, così come confermato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalle indagini epidemiologiche dell'Istituto superiore della sanità, costituisce un grave e drammatico problema sanitario e ambientale, a causa della continua esposizione della popolazione alla diossina presente nell'atmosfera e alla grande quantità di rifiuti presenti, fonte di contaminazione del suolo e delle falde acquifere. da trascurare anche le criticità creatisi nella gestione dei rifiuti che, in tale campo e in maniera esponenziale, ha fatto proliferare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Dal 2009, nell'ambito delle attività della Conferenza permanente regionale, è stata prevista presso la prefettura di Napoli l'istituzione di un tavolo permanente, alle cui riunioni, susseguitesi nel tempo, hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, di enti locali, associazioni e comitati. In tale contesto, non è mancata l'elaborazione di strategie di contrasto successivamente attuate da personale di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e polizie provinciali e locali. Sono stati intensificati, dunque, i servizi di controllo del territorio mediante la predisposizione di specifiche e mirate attività lungo le strade periferiche e nelle località in cui è stato rilevato il maggiore numero di sversamenti. Nella sola provincia di Caserta, sono stati individuati al momento 50 principi di incendio, 162 persone sono state tratte in arresto e 121 sono state denunciate per deposito incontrollato di rifiuti. In considerazione della tipologia e natura dei materiali dati alle fiamme con maggiore frequenza (pneumatici, scarti di lavorazione tessile e di attività agricola, materiali edili), si è provveduto a intensificare i controlli presso rivendite di pneumatici, al fine di verificare l'osservanza di eventuali ordinanze comunali di divieto di deposito esterno all'esercizio di tali prodotti e la corretta tenuta dei registri di carico e scarico. Analogamente, sono state intensificate le attività di controllo su aziende tessili e agricole. È stata richiesta anche una maggiore attività informativa e investigativa in ordine alle modalità adottate dalle aziende e dagli esercizi commerciali rispetto allo scarico dei rifiuti. Al fine di intervenire in modo significativo, l'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, designato con decreto del Ministero dell'interno del 26 novembre 2012, ha istituito una cabina di regia per l'attivazione, con l'intervento della Regione Campania, delle Province e delle prefetture di Napoli e Caserta, dell'ARPA Campania e delle ASL, delle attività amministrative di integrazione a corollario dell'azione di contrasto posta in essere dalle forze dell'ordine e dalle polizie locali delle province di Napoli e Caserta. Tra le più importanti iniziative intraprese per il contrasto del fenomeno degli incendi tossici in Campania, è da segnalare il patto per la terra dei fuochi, firmato a Napoli lo scorso 11 luglio, con il quale è stata predisposta una serie di misure, che vedono il coinvolgimento della Regione, delle prefetture, delle amministrazioni provinciali di Napoli e Caserta, dell'ANCI Campania, delle associazioni ambientaliste e di 57 Comuni. Tale patto, oltre a rafforzare i vincoli e gli impegni degli aderenti per affrontare un tema così delicato, tende a definire un sistema unitario di interventi dove si integrano misure di carattere strutturale e misure straordinarie, attività di contrasto alle condotte illecite e attività rivolte ad affrontare i nodi amministrativi delle competenze, dell'applicazione delle norme, della disponibilità di risorse umane e strumentali, che spesso rappresentano un ostacolo per il perseguimento del risultato. Economicamente, con il predetto patto la Regione Campania si è impegnata a stanziare, per le attività di controllo e di tutela ambientale, la somma di 5 milioni di euro, destinata a finanziare progetti presentati dagli enti firmatari per iniziative di videosorveglianza e telecontrollo di aree critiche e per l'acquisizione di infrastrutture e tecnologie avanzate, da assegnare agli operatori impegnati nelle specifiche attività di sorveglianza e antincendio. Il suddetto patto prevede, inoltre, in materia di trasparenza, sul sito *web* della prefettura di Napoli, il cosiddetto portale «Prometeo», costantemente aggiornato su tutti gli interventi e sulle misure di contrasto e di governo adottate dai Vigili del fuoco e da tutte le forze di polizia a contrasto del fenomeno. Tale strumento garantisce pertanto la circolarità del flusso informativo e la tempestiva individuazione dei fattori di crisi e delle aree sensibili. I dati finora inseriti segnalano oltre 1.700 pattugliamenti effettuati, 230 controlli su attività economiche, di cui 102 su rivenditori di pneumatici e 90 su attività produttive, 8 arresti), 37 denunce all'autorità giudiziaria, 270 contravvenzioni, 35 aree adibite a smaltimento illegale sottoposte a sequestro penale, 22 veicoli sequestrati adibiti a traffico illecito di rifiuti. Sono state inoltre individuate 22 attività economiche svolte in assenza di autorizzazione e in 29 casi sono emerse, nel corso dei controlli, situazioni di lavoro nero e irregolare. Sono state chiuse 7 aziende tessili illegali gestite da operatori economici di origine cinese. Sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 60.000 euro. Le statistiche dei Vigili del fuoco relative al periodo gennaio-maggio registrano, invece, per la provincia di Napoli, un calo significativo degli interventi di spegnimento, 653, rispetto ai corrispondenti periodi del 2012 e del 2011, quando furono 1.248 e 2.754. Anche la provincia di Caserta fa registrare, nell'analogo periodo, una contrazione, passando da 472 interventi nel 2012 a 212 nel 2013. Oltre alla trasparenza delle attività, il patto promuove, sotto diversi aspetti, forme di collaborazione e partecipazione aperte delle associazioni ambientaliste, chiamate a condividere il programma, senza tralasciare i cittadini, valorizzando così il rapporto di fiducia tra le istituzioni e la popolazione. A testimonianza della volontà degli enti locali, delle istituzioni e dei cittadini di impegnarsi concretamente nella lotta al fenomeno dell'incendio di rifiuti e della percezione diffusa dell'utilità e dell'efficacia degli strumenti di prevenzione e contrasto già messi in atto in questi mesi, numerose amministrazioni comunali delle province di Napoli e Caserta, non ricomprese tra quelle firmatarie del patto, in questi giorni stanno chiedendo di potervi aderire. A dimostrazione che il problema sia di particolare importanza e all'attenzione del Ministero dell'ambiente, vi è il fatto che proprio il Ministro dell'ambiente - come è stato ricordato anche dall'interpellante - a pochi giorni dal suo insediamento ha subito visitato la cosiddetta terra dei fuochi, per prendere diretto contatto con la realtà ambientale del territorio compreso tra la provincia di Napoli e Caserta, dove si verificano continui roghi di rifiuti, soprattutto di pneumatici usati e abbandonati. In particolare, è stato visitato il territorio di alcuni Comuni della provincia di Caserta, commissariati a causa delle infiltrazioni della criminalità organizzata, dove il problema della gestione illecita dei rifiuti presenta specifiche criticità.

e sono state apprezzate le iniziative e le attività avviate e in corso dei prefetti di Napoli e di Caserta e dell'incaricato dal Ministro dell'interno per contrastare l'illecito incenerimento dei rifiuti abbandonati. Successivamente a tale visita, al fine di contrastare il fenomeno dei roghi, in particolare di pneumatici, il Ministro si è impegnato a favorire un intervento coordinato tra i Comuni della provincia di Napoli e Caserta ed il consorzio per il riciclaggio dei pneumatici usati. Da qui, lo scorso 20 giugno il Ministero dell'ambiente, la Regione Campania, la prefettura di Napoli e di Caserta, il Comune di Napoli e di Caserta, l'incaricato dal Ministro dell'interno per il fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti in Campania e il consorzio per il riciclaggio dei pneumatici usati hanno stipulato un protocollo d'intesa «per l'attuazione di interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso abbandonati nel territorio delle province di Napoli e Caserta». Con tale protocollo, i Comuni di Napoli e Caserta, nonché gli eventuali altri Comuni interessati delle province di Napoli e Caserta, si sono impegnati, nell'ambito dell'espletamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, al fine di assicurarne una gestione corretta e scongiurare il continuo verificarsi di roghi, a rintracciare e raccogliere i pneumatici fuori uso abbandonati nei rispettivi territori e a conferirli presso idonei centri autorizzati. Poiché il predetto protocollo prevede la costituzione di un comitato di vigilanza, lo scorso 12 agosto il Ministero dell'ambiente ha richiesto ai firmatari dell'intesa la designazione dei componenti. Parallelamente, è stato perfezionato il decreto del Ministero dell'ambiente con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e di ripartizione delle disponibilità del fondo per la per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fondo, destinato al finanziamento di interventi di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e riciclaggio, è ripartito tra i Comuni delle Regioni oggetto di procedura di infrazione comunitaria o di condanna da parte della Corte di giustizia per violazione o non corretta applicazione delle direttive in materia di gestione dei rifiuti, i cui consigli comunali risultino sciolti con decreto del Presidente della Repubblica a causa di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso mafioso o similare, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza stabilito dall'allegato avviso. Tra i Comuni che possono essere beneficiari di tali finanziamenti rientrano anche quelli della Regione Campania. n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, è stato introdotto il divieto temporaneo di importazione

nel piano regionale, situazione che rende opportuno impedire che il peso dei rifiuti speciali e di quelli urbani pericolosi nella Regione sia aggravato dal carico di quelli importati. Non si può poi mancare di sottolineare le iniziative di rilievo e sollecitazione poste in essere dal Ministro dell'ambiente, onorevole Andrea Orlando, nei confronti dei vertici delle istituzioni partenopee volte al completamento delle iniziative regionali per la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, così come previsto nel Piano regionale, necessaria per migliorare la situazione ambientale regionale e per superare le contestazioni avanzate dalla Commissione europea nell'ambito di diverse procedure

dati sanitari ed ambientali del territori campani funzionale all'individuazione delle aree per le quali sono necessari ulteriori approfondimenti. Il percorso progettuale multidisciplinare (ambientale, epidemiologico, tossicologico) tenderà a verificare le possibili connessioni tra lo stato dell'ambiente e la salute dei cittadini. Con riferimento alla richiesta di deroga al patto di stabilità per gli interventi finalizzati alla rimozione dei rifiuti, pur riconoscendo il valore della proposta, occorre esprimere una certa prudenza, connessa al reperimento di adeguate risorse finanziarie a compensazione degli effetti peggiorativi che la stessa può determinare sui saldi di finanza pubblica. Da ultimo, vi è da evidenziare che i siti di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. L'individuazione dei siti di interesse nazionale avviene mediante decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate, ed elenca una serie di principi e criteri direttivi cui attenersi. In particolare, gli gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004; il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato; l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più Regioni. Alla luce di quanto anzidetto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della disciplina riportata, ha provveduto alla ricognizione Grazie, agro aversano non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 36-*bis* della legge n. 134 del 2012, pertanto non può rientrare tra quelli novellati come siti di interesse nazionale. Questo aspetto non esclude l'attenzione posta sull'area in oggetto ai fini dei dovuti interventi di tutela ambientale.

come rappresentanti istituzionali, abbiamo parlato con le forze dell'ordine locali che non sono a conoscenza di questa camera di regia, di corsi e di linee guida: sono persone che lavorano tutti i giorni a mani nude sul territorio, senza i mezzi e gli strumenti necessari. Se le parole che lei ha detto fossero state la presentazione

egli venga a dirmi qui, in faccia, che questa è soltanto una pantomima per tenere buoni i comitati. Ma quali comitati, quelli ufficiali? Quali sono i comitati che avete sentito? PRESIDENTE.

Ritengo, comunque, in via preliminare, e prima di rispondere ai quesiti posti, che a tali disposizioni vada comunque riconosciuto il merito di avere individuato strumenti che hanno consentito la messa in commercio di medicinali che, prima dell'entrata in vigore della medesima norma in Italia, non erano a disposizione dei pazienti neanche nella fascia C, cioè a pagamento, mentre - come è noto - potevano essere acquistati in altri Paesi dell'Unione europea. Le norme hanno impattato anche su medicinali che giustamente, lo ripeto, hanno suscitato grande interesse e aspettative, considerato che si è trattato dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali antitumorali. Come è evidente, fin dalla prima fase attuativa sono emerse difficoltà, connesse soprattutto alle diverse possibilità di accesso per i cittadini, attesi i costi significativi dei medicinali in questione e ai tempi italiani (ripeto, italiani) troppo lunghi rispetto agli altri Paesi europei per le procedure autorizzative di classificazione ai fini della rimborsabilità o meno dei medicinali. La problematica è stata oggetto, come è noto, anche di importanti sollecitazioni e iniziative di entrambi i rami del Parlamento, come l'interrogazione che discutiamo oggi. Per superare tali criticità e per rispondere positivamente alle richieste di tanti cittadini, impossibilitati per motivi economici ad accedere a tali medicinali, e per venire incontro alle forti sollecitazioni del Parlamento, il Governo, su proposta del ministro Lorenzin, ha presentato tempestivamente una norma per superare tutte le difficoltà emerse. Tale norma, che tra l'altro è stata anche perfezionata da emendamenti di iniziativa parlamentare, è stata approvata nel corso della conversione del cosiddetto decreto-legge del fare: ha prescritto il termine perentorio di 100 giorni per la conclusione dell'intera procedura autorizzativa da parte dell'AIFA e ha previsto anche misure sanzionatorie per garantire il rispetto dei medesimi tempi. Rassicuro, comunque, che è intenzione del Ministero vigilare affinché i tempi vengano rispettati, atteso l'impatto e l'urgenza delle finalità cui la norma è diretta. Per quanto riguarda la procedura per la classificazione dei medicinali, oggetto della interrogazione, comunico che, per il primo, si è dato avvio all'*iter* negoziale per la classificazione in fascia H ospedaliera ad oggi la procedura è in fase di valutazione da parte della commissione tecnico-scientifica; per il secondo, l'azienda produttrice ha già chiesto la classificazione in classe H ospedaliera, la domanda di negoziazione del prezzo è già all'esame della Commissione tecnico scientifica dal mese di luglio 2013 e sono ancora in corso approfondimenti. Dalle informazioni acquisite, e fatti salvi impedimenti che ad oggi non mi è dato di conoscere, ritengo che i tempi previsti per l'immissione in commercio saranno rispettati. Da ultimo, per quanto attiene al principio generale di accesso universale alle cure, quale punto di forza del Servizio sanitario nazionale, non posso che convenire su quanto segnalato dai senatori interroganti. Nel contempo però devo rilevare che tali criticità non riguardano solo l'ambito segnalato, ma hanno purtroppo una portata di carattere generale per tutta l'assistenza sanitaria.

e all'interno delle stesse e tentare, quindi, di garantire l'universalità di accesso alle cure, a sostegno del diritto alla salute costituzionalmente protetto.

di reti oncologiche regionali, che ragionino quindi in termini statistici qualitativi, e di diagnostiche uniformi, in modo tale da poter avere

Signor Presidente, con l'interrogazione all'ordine del giorno la senatrice Valentini chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere per garantire l'efficienza del servizio di soccorso dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Roma Al riguardo, voglio premettere che la situazione dei mezzi di soccorso presso il comando di Roma è in linea con quella riscontrabile sul resto del territorio nazionale. Pur registrandosi talune difficoltà nel rinnovo del parco automezzi a causa dell'attuale congiuntura economica, il comando dispone di oltre 70 mezzi operativi, dislocati presso la sede centrale e i distaccamenti. Nel corso dell'anno saranno acquisiti ulteriori mezzi, per la parziale sostituzione di quelli più vetusti. Il comando provinciale è costituito, oltre che dalla sede centrale, da 32 distaccamenti, nonché dai nuclei speciali sommozzatori e radioriparatori. La previsione organica relativa al personale operativo permanente (capi reparti, capi squadra e vigili) è di 1.640 unità. L'attuale dotazione, di 1.515 unità, fa registrare una carenza di circa l'8 per cento, peraltro in linea con il dato nazionale. Con tali unità operative, ripartite su 4 turni di servizio, viene assicurata la partecipazione, in media, di circa 265 vigili per turno. Dal punto di vista dell'equipaggiamento, pertanto, il comando di Roma risulta essere dotato di mezzi adeguati a svolgere quotidianamente i servizi d'istituto. Invero, negli ultimi cinque anni, sono stati svolti circa 50.000 interventi all'anno. Posso assicurare, quindi, che la sicurezza e l'incolumità pubblica costituisce la principale preoccupazione del Governo e del Ministero dell'interno e che, nonostante i vincoli non potranno essere compromessi i livelli di efficienza del sistema di soccorso che vede fortemente impegnato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con uno straordinario sforzo operativo. da ultimo ricordare che il Governo ha approvato due provvedimenti, il decreto sicurezza e il decreto conosciuto come D'Alia, che sostanzialmente recepisce istanze molto significative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra le misure più importanti, citerei l'assunzione di 1.000 nuovi vigili del fuoco e l'istituzione di un fondo per l'emergenza che va incontro

*(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, devo dire che ho seguito con molta attenzione la questione del comparto sicurezza, in particolare quella dei Vigili del fuoco

operando a favore del comparto dei Vigili del fuoco, che è un comparto delicatissimo e particolare che ha un grande bisogno di interventi urgenti e straordinari. Infatti, soprattutto in questi ultimi anni, in Italia e all'estero, è stato è stato protagonista di diversi scenari emergenziali e di complessità straordinarie nel nostro Paese. È un comparto, però, che ha tanti problemi.

dovere istituzionale di prendere atto di ciò che mi dice il Sottosegretario, che ha sicuramente informazioni più esatte delle mie. Quello che Grazie,

chiarimenti in merito alla paventata chiusura del distaccamento aeroportuale dei Vigili del fuoco a Parma, nonché circa la possibilità di procedere ad una razionalizzazione dei distaccamenti misti presenti in Provincia, con l'istituzione di un eventuale nuovo distaccamento a Fornovo di Taro. Si chiede, inoltre, di conoscere quali iniziative si intendano adottare per consentire la piena operatività delle dotazioni strumentali a disposizione del comando di Parma. Il comando dei Vigili del fuoco di Parma, oltre alla sede centrale, attualmente dispone di due distaccamenti permanenti: un distaccamento volontario e un distaccamento aeroportuale. L'organico teorico del relativo personale operativo permanente è di 208 unità. Attualmente le presenze sono pari a 219 unità, anche se risultano carenze nel personale qualificato (in particolare capi squadra e capi reparto), che si pensa tuttavia di colmare con il completamento dell'*iter* concorsuale dei passaggi di qualifica, previsto ormai per la fine di quest'anno. Allo stato attuale, non è prevista nessuna riduzione dì organico o modifica nelle sedi di servizio, né la cessazione dell'attività dei distaccamenti indicati. In particolare, la paventata chiusura del distaccamento aeroportuale non è attualmente ipotizzabile, essendo le attività del presidio strettamente connesse al dispositivo di soccorso dello scalo presso l'aeroporto di Parma. Riguardo, invece, alla possibile apertura di un'ulteriore sede distaccata a Fornovo di Taro, nonostante la nota condizione di indisponibilità delle risorse, sono stati avviati i necessari approfondimenti, tramite gli uffici territoriali del Corpo e gli enti locali, per l'individuazione di un'idonea sede di servizio. In merito, infine, alle dotazioni del comando di Parma, gli automezzi in servizio risultano sufficienti in relazione alle squadre presenti sul territorio e, quanto al loro stato d'uso, leggermente superiori alla media nazionale. I mezzi d'intervento per garantire l'assoluta sicurezza degli operatori e la massima efficacia nel soccorso sono soggetti a manutenzioni programmate, straordinarie e a controlli periodici, per cui, a rotazione, una percentuale dei mezzi viene posta temporaneamente fuori servizio. Solo per limitati periodi tre autopompe APS sono state poste fuori servizio, su un totale di undici in dotazione. Relativamente ai mezzi speciali a disposizione, un'autogru e un'autoscala risultano attualmente in manutenzione. Concludo ribadendo la costante attenzione del Ministero dell'interno affinché venga sempre garantito il regolare funzionamento delle dotazioni strumentali in uso e altresì assicurata la piena operatività dei presidi sul territorio.

sia la risposta in ordine alla sede del distaccamento dell'aeroporto di Parma, sia l'attenzione e lo studio in ordine all'apertura della sede di Fornovo

Per quanto riguarda la manutenzione della strumentazione, non posso scendere sul piano tecnico: mi rimetto, quindi, alle sue valutazioni, dalle quali emerge anche l'attenzione a che il livello di efficienza non venga diminuito, ma aumentato.